La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 25 novembre. È stato innanzitutto stabilito che le dichiarazioni di voto e il voto finale sul disegno di legge di riforma della professione forense avranno luogo martedì 23 novembre, a partire dalle ore 16,30. L'ordine del giorno della seduta pomeridiana odierna è stato integrato con i seguenti argomenti: Discussione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari al fine di sollevare conflitto di attribuzione su una questione concernente l'ex ministro Mastella. Esame del disegno di legge sull'esecuzione domiciliare di pene detentive, con ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Ratifiche di accordi internazionali. Il calendario di questa settimana prevede inoltre la discussione di mozioni, con la consueta ripartizione dei tempi, sui benefìci a favore di vittime del terrorismo, sulle candidature alle elezioni regionali e amministrative, nonché sulla patologia della depressione. La prossima settimana, nella seduta pomeridiana di martedì 23 novembre, oltre alle dichiarazioni di voto e alla votazione finale del disegno di legge di riforma della professione forense, come già ricordato, alle ore 19 la Presidenza comunicherà il proprio parere all'Assemblea sul contenuto del disegno di legge di stabilità. Nel corso delle predette dichiarazioni di voto, la 5a Commissione permanente è autorizzata a convocarsi per l'esame preliminare del disegno di legge di stabilità, ai fini dell'espressione del parere al Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Subito dopo la comunicazione del Presidente, ai sensi della richiamata norma regolamentare, saranno assegnati i documenti finanziari e avrà pertanto inizio la sessione di bilancio, i cui tempi saranno partitamente definiti dalla prossima Conferenza dei Capigruppo. Al riguardo, è stato sin d'ora stabilito che la prossima settimana si riuniranno le Commissioni permanenti in relazione ai rapporti da trasmettere alla Commissione bilancio. Quest'ultima concluderà i propri lavori in sede referente entro venerdì 3 dicembre. Nella settimana successiva i documenti finanziari saranno portati all'esame dell'Assemblea, affinché le votazioni finali avvengano entro venerdì 10 dicembre. Per quanto riguarda i lavori della prossima settimana, tenuto conto dell'impegno delle Commissioni sui documenti di bilancio, l'Assemblea terrà sedute, in orari contenuti, nelle giornate di mercoledì 24 e di giovedì 25 novembre per la discussione delle mozioni eventualmente non concluse entro la giornata di domani, nonché della mozione Scanu ed altri sul modello di difesa. Nel pomeriggio di domani e di giovedì 25 novembre avrà luogo il sindacato ispettivo. Nel corso della riunione i Capigruppo hanno anche affrontato il tema della verifica politica, in relazione alla quale il Presidente del Consiglio renderà comunicazioni al Senato lunedì 13 dicembre alle ore 9. La discussione generale si concluderà intorno alle ore 14. Le dichiarazioni di voto sulle proposte di risoluzione inizieranno martedì 14 dicembre alle ore 9. Seguiranno le operazioni di voto.

concernente l'applicazione della disciplina relativa ai reati ministeriali con riferimento a procedimenti penali pendenti nei suoi confronti presso il tribunale di Napoli***

davanti alla Corte costituzionale in ragione della violazione della competenza del Tribunale dei ministri che ha comportato l'omissione di quegli obblighi di autorizzazione o comunicazione che costituiscono la premessa indispensabile affinché il Senato possa compiere autonomamente la propria valutazione sulla qualificazione dei reati in questione. Chiedo al relatore, senatore Mercatali, se intende integrare la relazione scritta.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, come risulta dalla relazione del collega Mercatali (che - lo dico per chi ci ascolta attraverso la radio e la televisione - è un collega dell'opposizione, del Partito Democratico, nell'ambito di questo procedimento), la condotta che ha seguito la procura della Repubblica di Napoli deve considerarsi lesiva delle attribuzioni costituzionali del Senato, non avendo in alcun modo l'autorità giudiziaria rispettato quanto prevede la legge costituzionale gennaio 1989, n. 1. I procedimenti penali avviati nei confronti dell'onorevole Mastella si riferiscono infatti a fatti avvenuti nel periodo in cui egli rivestiva la carica di Ministro della giustizia, il pubblico ministero di Napoli ha ritenuto di non attivare la procedura prevista dalla legge costituzionale che prevede la competenza del cosiddetto tribunale dei ministri ai fini dello svolgimento delle indagini e delle conseguenti determinazioni in ordine alla richiesta di autorizzazione a procedere, ovvero all'archiviazione asistematica (come l'ha chiamata ultimamente la Corte costituzionale in una sentenza molto importante, la sentenza n. 241 del 2009 sul caso Matteoli). Quindi, sussistono per noi tutti i presupposti per sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale essendo state menomate, come dicevo, le nostre attribuzioni in materia. Il caso Matteoli e il caso Castelli sono già stati trattati dal Parlamento in questa legislatura: essi hanno molte analogie con il caso che trattiamo noi oggi in quest'Aula quest'Aula e hanno dimostrato come una parte dalla magistratura - per fortuna minoritaria - persegua un disegno contrastante con il principio di leale collaborazione tra le istituzioni e diretto a negare sistematicamente le attribuzioni costituzionalmente previste a favore del Parlamento, scendendo in campo per azzoppare degli avversari ideologicamente individuati. Come ho detto, questa interpretazione della disciplina costituzionale e legislativa in materia di reati ministeriali è già stata apertamente sconfessata e criticata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 241 del 2009 che, come pochi hanno notato, è una sentenza che ha visto la sostituzione del giudice relatore. Nella Corte il giudice relatore incaricato era il giudice De Siervo e la sentenza ha poi avuto come estensore il giudice costituzionale avvocato Frigo. In quella sentenza, la Corte ha chiarito quale debba essere il corretto bilanciamento tra i valori in gioco, che sono la funzione di governo, da una parte, e l'efficienza della funzione giudiziaria, Per noi si tratta di capire se la posizione di questa parte minoritaria della magistratura sia solo frutto di un'errata lettura delle norme, che dovrebbe essere essere ormai definitivamente tramontata dopo la sentenza della Corte, o se invece è espressione della pervicace volontà di condizionare la politica, alla faccia della proclamata distinzione fra potere giudiziario e potere

Concludo dicendo che il Presidente del Consiglio aveva proposto, poco tempo fa, la creazione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi nei quali le procure si sono trasformate in strumenti di lotta politica, la galleria degli orrori e della faziosità giudiziaria è ormai molto lunga. Probabilmente i casi Matteoli, Castelli e - adesso - Mastella fanno parte di questa galleria degli orrori giudiziari. Se fossimo un Paese normale, quella Commissione parlamentare di inchiesta sarebbe già stata istituita, perché è interesse - ripeto: se fossimo un Paese normale - di tutte le parti politiche chiarire definitivamente se esiste, come purtroppo esiste, una parte della magistratura che agisce per altri fini, diversi da quelli istituzionali della magistratura. Noi non siamo però un Paese normale e, dunque, per la Commissione di inchiesta aspettiamo la XVII legislatura.

esprimo condivisione rispetto alla relazione della Giunta che, sia pure sinteticamente, ha espresso le valutazioni che il caso particolare richiedeva, ribadendo in questa circostanza soltanto alcuni rilievi in ordine alle tante anomalie che hanno contraddistinto questa vicenda. Come ricordava poco fa il senatore Mazzatorta, ci sono state ben tre richieste inoltrate e rimaste inevase, che hanno di fatto rallentato anche i tempi della Giunta per potersi pronunciare.

ritengo che lo stesso provvedimento con il quale il Gup di Napoli, sostanzialmente condividendo la posizione del pubblico ministero, ha tentato di fornire una giustificazione all'operato della magistratura inquirente, costituisca una pronuncia dalla portata per così dire eversiva: si pretende infatti di ribaltare il sistema delle garanzie costituzionali con un ordine argomentativo che è che è sostanzialmente contraddetto non solo dal dato normativo, dall'articolo 96 della Costituzione e ancor più dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, ma anche dalla recente pronuncia della Corte costituzionale, la n. 241 del 2009, che, in maniera molto chiara, con portata scultorea, ha definito i margini che distinguono i rapporti tra l'autorità giudiziaria ed il Parlamento nell'esame, in particolar modo, delle fattispecie dei reati ministeriali.

delle determinazioni assunte in merito alla vicenda processuale dell'allora senatore Mastella - nella sua qualità di Ministro, beninteso - hanno fortemente leso quel diritto che la Corte costituzionale ha definito come costituzionalmente protetto del Parlamento ad essere informato. sia perché spetta al Parlamento, come accade nel dibattito di oggi, di poter esaminare la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione, non condividendo l'operato dell'autorità giudiziaria che ha omesso una serie di adempimenti necessari, e quindi ha impedito al Senato di potersi pronunciare sulla ministerialità stessa del reato, sia soprattutto perché, attraverso il coinvolgimento diretto del Parlamento, in ossequio anche al principio di economicità dei procedimenti, si evita che il Senato sia costretto, a pronuncia definitiva intervenuta, a dover sollevare in quella sede il conflitto. In caso, con altissima probabilità di successo, di una pronuncia favorevole della Corte costituzionale, si azzererebbe quindi l'intero procedimento e tutti gli atti che sono stati compiuti, ricominciando daccapo, con tutti gli effetti che ne derivano anche sotto il profilo della lesione dei diritti del singolo e soprattutto del diritto del Parlamento ad avere piena titolarità nel procedimento che precede la pronuncia. Rispetto alla relazione della Giunta, osservo, anche richiamando il precedente deliberato di quest'Aula relativo alla vicenda del senatore Castelli, che comunque, secondo una lettura anche più ampia del dettato costituzionale, è la stessa qualificazione del reato in termini di ministerialità, o meglio la valutazione definitiva sulla qualificabilità del reato in termini ministeriali, che spetta a questa Assemblea; naturalmente questa anomala, irrituale e, possiamo definirla tranquillamente così illegittima procedura che ha contraddistinto la vicenda del senatore Mastella ha di fatto leso anche questa prerogativa del Parlamento. Sicché, rispetto alle conclusioni rassegnate dalla Giunta, non possiamo che confermare in questa sede la nostra piena condivisione e una convinta adesione alla decisione di sollevare conflitto di attribuzione.

in questo caso sia le considerazioni sia le valutazioni che abbiamo fatto in Giunta, che hanno trovato una convergenza unanime di tutti i componenti di questa, non si prestino ad interpretazioni di vario tipo e di varia natura. Abbiamo seguito un ragionamento lineare e un riferimento giuridico puntuale alle leggi alle quali ci siamo appellati e siamo giunti a questa conclusione in maniera unanime. A maggior ragione, ribadisco quella relazione e quei contenuti. Mi limito a questo, anche perché, se

Presidente, onorevoli colleghi, bisognerà fare un po' di chiarezza, dal momento che sono stati evocati dei precedenti in modo del tutto improprio. Il senatore Mazzatorta evocava in quest'Aula il precedente che riguardava l'ex ministro Castelli. Voi ricorderete, colleghi, che in quella vicenda si trattava di decidere sulla ministerialità di un fatto.

All'epoca, il problema era se il saltellare scandendo il ritornello «chi non salta italiano è» rientrasse nelle prerogative ministeriali, con tutti gli annessi. Si citò nel caso la non remota ipotesi in cui il ministro Castelli, ritornando in terra dal suo saltello, avesse involontariamente colpito un ignaro passante provocandogli una lesione colposa. Il problema era

che saltellare cantando «chi non salta italiano è» era reato ministeriale. Qui stiamo invece esaminando un'altra questione, questione, cioè che quest'Aula non sia stata messa in condizione di pronunziarsi sulla ministerialità o meno di un reato. Dunque l'evocazione dei precedenti è stata abbastanza impropria. La risposta è di natura tecnico-giuridica ed è stata condensata in maniera, a mio parere, inoppugnabile e non criticabile, dal punto di vista tecnico, dal relatore Mercatali.

il problema del conflitto di attribuzione. Questa attività deve essere infatti finalizzata al ripristino del corretto svolgimento del processo, secondo le indicazioni della legge e della nostra Carta

sentito succintamente esposta dal senatore Mercatali, hanno ritenuto che sia necessario sollevare il conflitto di attribuzione per vedere rispettata la legge costituzionale n. 1 del 1989. Mi potrei fermare qui. È un procedimento abbastanza anomalo quello che abbiamo avuto la possibilità di esaminare, anche perché, a differenza di quanto ho sentito dire dal senatore Mazzatorta, il ritardo nella trasmissione degli atti al Senato non è derivante da una iniziativa di rallentamento dell'autorità giudiziaria, ma dal fatto che, come ci ha raccontato per iscritto l'allora ministro Mastella, semplicemente il Ministero della giustizia si era dimenticato per un anno di rispondere alle sollecitazioni del Presidente del Senato. Solamente lo scorso 4 ottobre ha inoltrato all'autorità giudiziaria la richiesta di avere le carte del procedimento. Abbiamo lavorato su produzioni di parte certificate dal tribunale di Napoli. Ci sentiamo di poter assumere questa decisione in tutta serenità ed in tutta coscienza, senza ovviamente quelle alterazioni del tutto ideologiche che abbiamo sentito nell'argomentazione e nella motivazione di alcuni colleghi che mi hanno preceduto. Direi anzi che queste sono contrarie alla causa che il Senato va a proporre alla Corte costituzionale: un migliore *aplomb*, una ulteriore serenità, una maggiore asetticità delle nostre posizioni gioverebbe senz'altro alla prospettazione delle ragioni di questa Camera, e facciamo voto nel senso che tutte le altre ragioni di tipo ideologico siano espunte dalla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica.

affinché il Senato promuova conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale con riguardo alla richiesta inoltrata dall'onorevole Mastella. **È approvata.** La

è presente in Aula una delegazione di studenti della scuola media «Pietro Tacchi Venturi» di San Severino Marche, in Provincia di Macerata, cui va il saluto dell'Assemblea.

e che viene riproposto oggi all'Aula del Senato nell'identico testo al fine di agevolarne il più possibile la rapida entrata in vigore.

per tutti i detenuti con pena residua uguale o inferiore ad un anno la possibilità di scontare la suddetta pena residua presso la propria abitazione o presso altro luogo ritenuto idoneo,

viene modificato l'articolo 385 del codice penale al fine di aumentare in modo sostanziale la pena della reclusione per chi si rende responsabile del delitto di evasione. All'articolo 3, viene introdotta una nuova circostanza aggravante per chi abbia commesso il fatto in particolare, un delitto non colposo - durante il periodo in cui era stato ammesso a una misura alternativa alla detenzione. L'articolo 4, inoltre, reca disposizioni che mirano a rendere disponibili risorse per provvedere all'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, e in particolare all'assunzione di quasi 2.000 nuovi agenti di polizia penitenziaria. In sostanza, si tratta di un disegno di legge che mira a far fronte alla situazione di emergenza nella quale si trovano le carceri italiane, da un lato appunto, a circa 7.000 detenuti di espiare questo residuo di pena al di fuori delle carceri, dall'altro rendendo disponibile al più presto quasi 2.000 nuovi agenti di polizia penitenziaria per far fronte Grazie,

Signor Presidente, come ho avuto modo di dire in diverse occasioni lo stato dalle carceri nel nostro Paese è gravissimo e rappresenta una vera e propria emergenza umanitaria. Secondo le stime di «Ristretti Orizzonti» quasi uno su due degli oltre 63.000 detenuti risulta in attesa di giudizio e ben 19.558 sono i detenuti condannati con pena residua inferiore a tre anni, mentre quelli con pena residua inferiore a un anno sono 3.214.

Il tasso complessivo di sovraffollamento è dunque pari al 146 per cento, mentre il personale di polizia si ferma ad appena l'86,2 per cento dell'organico previsto, che in altri termini vuol dire che manca all'appello il 13,8 per cento delle forze ritenute necessarie. I primi mesi del 2009 hanno fatto registrare un triste primato rispetto agli ultimi anni: sono stati 28 i casi di suicidio nelle carceri;

Il dato parziale è il più elevato registrato ad oggi dal 2002, anno in cui è stato pubblicato il primo rapporto sui suicidi in carcere, e va di pari passo con l'aggravamento del sovraffollamento delle carceri; e meno male che la nostra Costituzione, con grande civiltà, non prevede la pena di morte. Secondo il Coordinamento nazionale degli operatori per la salute nelle carceri italiane, quasi la metà delle persone che scontano una condanna nei penitenziari italiani è costituita da tossicodipendenti o appartenenti all'eterogenea area dei consumi di sostanze stupefacenti, molto spesso non diagnosticati. Proprio il fatto di sottostimare il numero complessivo di pazienti porta a ipotizzare che durante tutto il corso dell'anno ci sia un numero di ingressi di tossicodipendenti pari a circa 50.000 persone, un fenomeno che viene registrato dagli operatori sanitari ma non dalle statistiche ufficiali. Per quanto riguarda i bambini in carcere, secondo i dati del Dipartimento di amministrazione penitenziaria riferiti al 30 giugno 2008, gli asili nido funzionanti nelle strutture carcerarie italiane sono 16. Sono 58 le detenute madri con figli che vivono con loro in istituto, quindi sono 58 i bambini minori di tre anni che trascorrono la loro vita in istituto. Basterebbero questi dati per mettere in evidenza lo stato delle nostre carceri: inaccettabile promiscuità e sovraffollamento, condizioni disumane, morti,

detenuti più giovani, un vero e proprio luogo di perdizione civile e morale che tende a confermare i reclusi come potenziali criminali e favorisce il loro reclutamento nelle file della delinquenza. Nessuno di noi pensa al carcere come a un luogo di vacanza dove si viva a spese dello Stato, ma è evidente che nel nostro Paese quella del carcerato è oggi una condizione non solo umanamente penosa e civilmente inaccettabile, ma anche socialmente onerosa perché non è utile a contrastare la tendenza a delinquere; anzi la favorisce. Paradossalmente, potremmo dire che nelle carceri italiane, nella situazione attuale, a spese dei contribuenti e della loro sicurezza, si creano e si formano le nuove leve della piccola e grande delinquenza. Paradossalmente possiamo affermare che molti dei nostri istituti penitenziari sono ormai fuori legge. Con questa legge potremo fare un piccolo passo avanti per migliorare lo stato delle cose, ma occorre modificarla, trarla fuori dalla logica dell'emergenza, trasformandola in un procedimento inteso come primo piccolo passo per avviare una fase nuova. Un passo al quale dovrebbe seguire, oltre l'emergenza, un generale reinquadramento del sistema carcerario,

giustizia nel nostro Paese, che sono ben altro dai lodi, dalle sospensioni dei processi per le alte cariche dello Stato e dai bavagli alla stampa. Abbiamo assoluto bisogno di avviare una fase nuova che che preveda non più rinviabili interventi strutturali senza i quali non sarà mai possibile approdare a un normale quadro di civiltà carceraria e giuridica, ma soprattutto una fase dove tutta una serie di pene possano essere scontate in modo diverso, dove al centro del sistema venga posto, insieme alla giusta pena, anche il possibile percorso riabilitativo, accentuando in tal senso l'attenzione soprattutto verso i detenuti più giovani e tentando così di spezzare quel malefico circolo che induce inesorabilmente a tornare a delinquere. Qui, signor Presidente, le chiedo veramente un momento di attenzione e di silenzio perché voglio dire con forza questa cosa. Voglio fare una raccomandazione a tutti noi, a tutti noi, alla stampa e ai *media*: non chiamate, per favore, questo decreto lo «svuota carceri». Il carcere non è un cestino da svuotare; i detenuti non sono rifiuti dei quali è urgente lo smaltimento. *(Applausi dai Gruppi* *PD e PdL)*. Sono esseri umani dei quali ci dobbiamo occupare con civiltà, con umanità e con la dovuta *pietas*, sia essa religiosa che laica.

È un tentativo di venire incontro al gravissimo problema del sovraffollamento carcerario prevedendo che le pene sino a 12 mesi vengano scontate presso il proprio domicilio. Noi sappiamo benissimo che questa previsione già esisteva nel nostro codice: è prevista la possibilità di scontare nel proprio domicilio le pene al di sotto di un certo limite. Cosa cambia rispetto alla normativa attualmente vigente? Cambia che per la pronunzia a regime ordinario è necessario un provvedimento del tribunale di sorveglianza. In genere, il detenuto con pena inferiore al limite previsto e titolare della possibilità di chiedere la detenzione domiciliare rivolge istanza. Da quel momento passano circa sei-sette mesi prima della decisione, sicché, quando interviene la decisione, di fatto l'anno è già scaduto.

sottoposta ad una verifica, non più del tribunale, ma del giudice di sorveglianza, ossia non più di un organo collegiale (che rende molto più complessa ovviamente la procedura) ma del singolo magistrato.

Era la soluzione più logica: s'interveniva su una norma del codice di procedura penale e si cambiava la competenza. Si è voluta seguire invece questa strada. Non ne siamo particolarmente entusiasti, perché l'automatismo creerà indubbiamente una serie di problemi

sottodimensionato rispetto all'onere del gravosissimo lavoro ad esso richiesto. Mancano 7.000 unità:

drammaticamente al collasso, e si va a fare pure un sondaggio! Diciamo che su questo fronte, dopo il quinto annuncio da parte del Ministro della giustizia

ci adegueremo quasi incoerenza.

di più - che, seguendo l'esempio da sempre portato avanti dai radicali in Parlamento, cominciano a visitare con cadenza mensile le carceri, ma lo dice la Corte europea dei diritti umani. Le nostre carceri, dal punto di vista della capienza regolamentare, dovrebbero consentire

di servizio prestato dal personale sanitario, per non parlare della totale assenza di educatori, psicologi o psichiatri. Questi sono i numeri di uno scandalo

da un organo collegiale alla decisione di un magistrato di sorveglianza, che quindi non necessariamente avrà i tempi, come ricordava il senatore Li Gotti,

ovunque si sieda oggi in quest'Aula, si sta portando avanti una politica che non può essere limitata alla costruzione di nuovi istituti o all'adozione di misure come queste, che letteralmente vanno contro la nostra Costituzione.

nonché una mozione approvata e firmata ‑ non li ho contati, ma credo siano un centinaio - da senatori di tutta la sinistra la quale, in uno dei punti qualificanti, chiedeva l'applicazione della detenzione domiciliare quale strumento centrale dell'esecuzione della pena relativa alle condanne di minore gravità. Oggi stiamo dando attuazione ad una

dalle 800 alle 1.000 unità. Dovremmo dire che molti stranieri finiscono in carcere, domanda alla quale dobbiamo anche saper dare un qualche tipo di risposta. Non si vivrà in modo

la capacità di prendere i responsabili dei reati - occorre dimostrarne la responsabilità, arrivare ad una condanna

Siamo convinti che per la questione del sovraffollamento la linea sia quella che è stata illustrata dal Ministro, cioè quei 47 padiglioni e quei 22.000 nuovi posti da realizzare. Però siamo anche convinti che

dove riuscire ad ottenere quantomeno di far scontare le pene anche in questo caso in modo più umano, più vicino al sistema parentale, più in grado di offrire assistenza di tutti i tipi a questi detenuti, ma nei Paesi d'origine. Ricordiamo che i costi per detenuto in questo Paese si aggirano sui 400-450 euro al giorno: proviamo a pensare qual è la cifra che riusciamo a dare in un mese ai nostri pensionati, che magari hanno lavorato una vita non proprio del tutto regolarizzata, con contributi non del tutto regolarizzati, eccetera. Il messaggio che vorremmo dare è che la Lega sa essere dura quando serve essere duri, ma sa anche essere comprensiva o morbida quando si deve essere tali. Abbiamo appena presentato un testo per inasprire

severo di sicurezza, tutte le altre persone tutto sommato possano rientrare in quell'altro alveo dell'umanizzazione della pena e che, a fianco degli altri modi di scontare le pene che conosciamo (affidamento ai servizi

consente in ogni caso di uscire, ma permette di rimanere in un ambito più umano, che sembra sia quello che anche i radicali e tutta la sinistra continuano a reclamare. L'unica cosa che vorremmo far presente al Governo Grazie, vorremmo che questo beneficio-sconto di pena fosse una specie di merito, cioè che a chi in carcere si comporta bene possa essere consentito anche di scontare 12 mesi presso il proprio domicilio, agli arresti domiciliari. Ma queste relazioni sulla condotta del detenuto che devono essere fatte dai direttori degli istituti penitenziari vorremmo che fossero oggetto di vigilanza e magari di supervisione, in modo che siano serie e che non siano sistemi fotocopia (arrivati agli ultimi 12 mesi, allora sì che scadremmo magari nella «svuota carceri») o che fosse per tutti

nonostante in linea di massima abbia perseguito altre politiche. Credo sia noto a tutti che da una decina d'anni a questa parte, forse anche di più, i detenuti sono andati via via aumentando. via aumentando. Quando il Parlamento fu costretto a dare un indulto di tre anni (era la prima volta che si verificava), vi era una situazione che poteva diventare esplosiva: vi erano 62.000 detenuti quando è stato pronunciato l'indulto. Adesso sono oltre 68.000, e ci avviamo ad arrivare a 70.000. Quindi, il problema attuale, signor Presidente e colleghi senatori, sta diventando di ordine pubblico,

trovino in carcere, quando è previsto che le nostre carceri possano contenere solo 43.000 detenuti. se vogliamo effettivamente continuare a fare una politica, che non è politica, di navigazione a vista, giorno per giorno, e con la demagogia, io credo che i problemi non si risolveranno. Signori della Lega Nord - e parlo a voi direttamente perché voi avete impostato la vostra politica sulla sicurezza, dimenticando altre - bisogna cominciare a vedere il problema nella sua complessità e con scadenze molto lontane.

modo di pensare e cominciamo a fare politica o, effettivamente, ci troveremo progressivamente ad affrontare questa situazione. Del resto, è dalla è dalla fine della guerra ad oggi che ogni quattro anni, mediamente, abbiamo avuto un provvedimento di amnistia o di indulto, proprio per questa ragione, cioè per il sovraffollamento delle carceri. A nulla è servita l'esperienza,

il quale ha riferito che i detenuti con pena inferiore ad un anno sono attualmente 11.000 e, di questi, dovrebbero uscirne, in quanto hanno un domicilio accettabile, 8.000. se si parla, invece, con i giudici di sorveglianza. Infatti, è vero che noi abbiamo trasferito la competenza dal tribunale ai giudici di sorveglianza; ma è altrettanto vero che questi giudici di sorveglianza hanno

allora ricordare ai colleghi della Lega Nord che l'aumento che c'è stato negli ultimi anni è stato dovuto, (oltre che al fatto che si è continuato a penalizzare illeciti,

se si trattava di recidivi che commettevano altro reato. Questa è stata una delle ragioni che ha fatto schizzare in alto il numero dei detenuti, perché se vengono diminuite le misure alternative al carcere è evidente che si hanno

si dimentica anche che, per motivi demagogici, con la legge Bossi-Fini condanniamo da uno a quattro anni, con arresto obbligatorio in flagranza di reato, chi non si è allontanato dal

*(PD)*. Vogliamo effettivamente svuotare le carceri? Cominciamo ad abrogare una disposizione del genere. Aveva ragione il senatore Divina quando diceva che noi paghiamo eccessivamente per ogni detenuto: ma vi siete mai chiesti se, invece di pagare

penitenziaria. In questo modo non si fa politica e non si andrà avanti in questo Paese.

denuncia da anni una assurda realtà: da lavoratori nelle strutture penitenziarie, gli agenti di Polizia penitenziaria si sono trasformati essi stessi in detenuti

lo sapete, e siete coscienti e consapevoli di quello che state facendo. Sono diventati prigionieri di uno Stato che non riesce ad affrontare i tre problemi principali che li affliggono: il sottorganico cronico, quello che stiamo affrontando in questo momento; i trattamenti economici inadeguati per il lavoro usurante e ad alto rischio; la mancanza di tutele penali e amministrative per reati commessi dagli agenti nel caso in cui questi siano determinati non da loro inadempienze ma proprio dalla mancanza di personale. Per non parlare dei suicidi del personale penitenziario, che state sottovalutando. Partiamo dall'organico. L'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame prevede che le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia siano destinate anche alla finalità dell'adeguamento dell'organico del Corpo di Polizia penitenziaria per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. La disposizione autorizza il Ministro ad assumere personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di Polizia penitenziaria, nei soli limiti consentiti dalle risorse derivanti dall'attuazione del richiamato comma. Caro Governo: si decide l'assunzione di 1.800 unità;

assunti! Infatti, la Ragioneria generale dello Stato in ben due occasioni ha restituito la relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia con la dicitura: «negativamente verificata». Vorrei

ma le dimentica il giorno dopo - questa norma potrebbe essere l'ennesima beffa, poiché i concorsi potrebbero essere banditi, gli agenti assunti, ma dopo un anno potrebbero finire i soldi per pagargli gli stipendi!

che nello stesso periodo si stima che andranno in pensione almeno 2.400 unità di polizia penitenziaria. Diamo allora i dati veri, non quelli fantasiosi. Spero di essere smentito, anzi me lo auguro: ma per risolvere la gravissima scopertura di uomini della Polizia penitenziaria, senza tenere conto dei pensionamenti, non bastano i 1.600 agenti, che forse potranno essere assunti, forse no;

Questa carenza di organico, si badi bene, non soltanto comporta dei gravi disagi per gli agenti, costretti a doppi turni e a straordinari non retribuiti, non soltanto inficia la sicurezza delle carceri, dove le porte fra le sezioni, come dicevo, devono rimanere aperte,

Devono esserci loro. Ecco perché la gravissima carenza organica ha tre risvolti drammatici: priva gli agenti di Polizia penitenziaria del diritto ad un lavoro umano; priva i detenuti dei diritti fondamentali (salute e rieducazione e contatti familiari); priva i cittadini della sicurezza. Se davvero il Governo vuole aprire nuovi padiglioni delle carceri

E allora, non si può continuare a fare promesse e non mantenerle. La condizione della Polizia penitenziaria non può essere una prigionia nella prigionia. Senza un impegno del Governo, la sicurezza sarà negata, la giustizia sarà per pochi e la pace sociale rimarrà un miraggio. Noi dell'Italia dei Valori siamo al fianco degli agenti che siedono in dal dottor Capece a tutti i sindacati di Polizia penitenziaria che stanno ascoltando, per rendere queste parole (sicurezza, giustizia e pace sociale) una realtà concreta. Chiediamo pertanto al Governo di fare altrettanto.

noi siamo assolutamente consapevoli del disagio in cui vive la Polizia penitenziaria, tant'è vero che alla Camera ci siamo battuti perché venisse introdotta nel testo del disegno di legge la previsione dell'aumento di organico e soprattutto dell'assunzione di personale di Polizia penitenziaria. Con un apposito ordine del giorno che sarà illustrato successivamente dal senatore Carofiglio, tra l'altro noi chiediamo anche che sia data

mi pare sufficientemente illustrato dal senatore D'Ambrosio - bensì l'ordine del giorno G101. Vorrei mettere in luce allora, signor Presidente, che la realtà della situazione carceraria italiana

psicologica a causa della cronica carenza di personale educativo; la pianta organica ministeriale prevede 1.331 educatori e 1.507 assistenti sociali, mentre in servizio al primo settembre risultavano 1.031 educatori e 1.105 assistenti sociali ossia circa 1 operatore ogni sessanta detenuti per un provvedimento, come quello in esame, che punta sulla deflazione carceraria per il miglioramento delle condizioni di vita negli istituti

che è decisivo per l'effettiva attuazione del provvedimento in esame. Dico questo perché l'articolo 1, comma 4, del disegno di legge enuncia che il magistrato di sorveglianza decide sull'applicazione della misura sulla base delle relazioni che riceve dalla direzione dell'istituto penitenziario sulla condotta tenuta dal detenuto durante la reclusione. In base alla normativa penitenziaria e nei fatti è l'educatore colui che osserva il comportamento del detenuto e provvede alla stesura della relazione di cui si servirà il magistrato di sorveglianza per decidere sulla misura alternativa. La strutturale carenza di educatori può determinare la redazione di un numero ridotto di relazioni da inviare al magistrato di sorveglianza, comportando di conseguenza un rallentamento della concessione di misure alternative. Si richiede quindi un impegno del Governo a sostenere e ad adottare iniziative idonee, tenendo presente che, oltre all'adeguamento della pianta organica corrispondente alla crescita della popolazione carceraria alla predisposizione di un piano straordinario di assunzioni di educatori penitenziari da attingersi dalla vigente graduatoria del concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di Educatore, Area C, posizione economica C1) che è stato indetto il 21 novembre 2003 e che non ha avuto seguito. Questo è un punto; ma vorrei mettere in luce anche un altro aspetto.

Noi dobbiamo considerare quale possibilità avrà la magistratura di sorveglianza, tenendo conto dello scarso organico della stessa (204: presenza 178)

subirà un forte impatto e soprattutto dovrà sostenerlo senza le risorse adeguate perché alla magistratura di sorveglianza manca non soltanto la presenza in organico di tutti i magistrati ma soprattutto la presenza

alimenta molte speranze nei detenuti e che può costituire un rischio di rivolta della popolazione carceraria, che sarà tradita nelle aspettative, impegna il Governo a prendere tutti i provvedimenti necessari perché la situazione sia adeguatamente supportata sotto il profilo dei magistrati,

Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G102, ma prima di arrivare al merito di questo atto desidero desidero sinteticamente illustrare quella che è la condizione delle carceri viste da chi, come me, esercita la funzione di garante dei diritti dei detenuti. La sensazione che ho quando ascolto un dibattito come quello di questa sera è che ci sia una conoscenza a macchia di leopardo del fenomeno carcerario,

quadri; di visite specialistiche rinviate di sei mesi in sei mesi; di interventi chirurgici non compiuti; di reclusi del peso di oltre 200 chili che compiono le loro funzioni fisiologiche in piedi perché non riescono ad entrare nei locali appositi. Parliamo di 55 suicidi di detenuti, ma anche di suicidi, lo diceva poc'anzi qualche collega, di guardie e anche di omicidi tra appartenenti alla Parliamo di alti dirigenti che si sono suicidati, parliamo di un costo giornaliero della reclusione che va da 120 a 250 euro. Parliamo di sprechi, come l'utilizzazione di un numero che varia da 6 a 12 agenti per custodire un recluso che deve subire un intervento chirurgico, perché non tutte le Province sono dotate di almeno un ospedale ove sia possibile ospitare, in reparti appositi, reclusi che devono subire un intervento chirurgico o effettuare altre cure ospedaliere. Stiamo parlando di un'Amministrazione penitenziaria forse esageratamente autoreferenziale, nel momento in cui affronta il tema di cui dovrebbe occuparsi, cioè l'organizzazione delle carceri. Parliamo ovviamente, inoltre, situazione insostenibile, anzi illegittima, illegale, come più volte l'Unione europea ci ha detto, condannandoci. Parliamo di una situazione di organico del personale della Polizia penitenziaria abbondantemente inferiore rispetto a quella che dovrebbe essere, ma parliamo pure di sprechi di personale della Polizia penitenziaria, che fa da scorta a persone che forse potrebbero avvalersi di altro tipo di tutela, o che lavora presso i bar delle carceri, quando invece potrebbe lavorare presso i diversi bracci, o che viene impiegato per funzioni di dattilografia o assistenza mentre forse farebbe meglio ad occuparsi di reclusi. Insomma, è una situazione che non può certamente essere affrontata a spizzichi e bocconi e che merita un ragionamento complessivo, in cui le parti in causa, e cioè la magistratura di sorveglianza, il Ministero della giustizia, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, le organizzazioni sindacali del personale della Polizia penitenziaria, e comunque dei dipendenti dell'amministrazione penitenziaria, la sanità penitenziaria, insomma tutti i soggetti che in qualche modo hanno a che vedere con il mondo delle carceri, svestendosi dei giudizi e dei pregiudizi che qualcuno di essi porta con sé e sedendosi attorno ad un tavolo, potrebbero costruire un modello di politica penitenziaria che raggiunga due obiettivi importanti. Il primo è il contenimento dei costi, oggi esageratamente lievitati a causa di una politica penitenziaria non sempre adeguata alla situazione che stiamo affrontando; il dovrebbe essere esattamente il contrario), è il pieno rispetto dell'articolo 27 della Costituzione, la dove si parla di rieducazione, di reinserimento. Ma il tema che stiamo affrontando non è recente. Alcuni degli spunti di questo intervento li ho tratti da un intervento dell'onorevole Maria Nicotra Fiorini nel 1953: ho utilizzato in alcuni passaggi di questo mio intervento le stesse sue parole. La verità è che di carceri non ne vuole parlare nessuno, perché ciascuno di noi forse pensa che il carcere costituisca l'aspetto terminale di un fenomeno di devianza sociale; invece è solo un aspetto transitorio. Il carcere è una fase della vita di chi commette un reato; ma chi commette un reato ha un prima, un durante e un dopo la pena: se non affrontiamo complessivamente questo circuito di natura criminale e post‑criminale, probabilmente non ne usciremo mai

il risparmio nel fenomeno delle traduzioni legate alle testimonianze dei detenuti. Il costo di una traduzione, soprattutto quando questa avviene con mezzi aerei, è notevolissimo e l'impiego di personale è cospicuo. Consentire l'acquisizione delle testimonianze attraverso la videoconferenza, come già accade, per esempio, nel caso di regime di 41-*bis*, potrebbe permettere all'amministrazione penitenziaria di risparmiare uomini, mezzi e risorse. Il secondo punto dell'ordine del giorno riguarda la possibilità per i reclusi di utilizzare più proficuamente il tempo di detenzione venendo essi autorizzati, attraverso un apposito provvedimento che il Governo potrebbe adottare, a svolgere corsi professionale non limitatamente a sei ore al giorno, ma estendendo estendendo la possibilità di partecipare a corsi per 12 ore al giorno. Peraltro, risulta ovvia la disponibilità di tempo di un recluso.

onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, da sempre molto sensibile alle tematiche dei reclusi - di questo le do atto - il Governo ha fatto molto per la politica penitenziaria del nostro Paese. Ha fatto molto con il piano carceri, con l'integrazione del personale della Polizia penitenziaria e l'impegno alla relativa assunzione. Ha fatto molto con questo provvedimento che, in parte,

Senatore Divina, ho ascoltato il suo intervento, e in parte lo condivido. Non è vero però che il carcere serva sempre: in alcuni casi non servirebbe affatto. Le faccio un esempio, e con questo concludo. Qualche settimana fa, andando a visitare il carcere dell'Ucciardone, vi ho trovato recluso un palermitano che era stato arrestato perché sorpreso a gettare masserizie per le strade di Palermo. È sbagliato gettare masserizie per le strade di una città, ma forse, se quel cittadino fosse stato condannato a pulire le strade della sua città che stava sporcando, l'effetto della pena sarebbe stato molto

passione, se non quella per risolvere il problema. Credo che un passaggio importante sia quello di costituire un tavolo attorno al quale senza pregiudizi si possa realizzare una politica penitenziaria che affronti i diversi aspetti, puntando al rispetto dell'articolo 27 della Costituzione e, quindi, pensando che dopo il carcere c'è comunque il reinserimento nella società. Se il carcere è stato utile, il reinserimento sarà produttivo, proficuo

dall'altra il contenimento dei costi dell'Amministrazione penitenziaria, raggiungibile con una più accorta politica dell'organizzazione nel suo complesso. Onorevoli colleghi, sarebbe in uno Stato, non rispettandosi i diritti dei detenuti e non costruendosi un sistema penitenziario adeguato a

questo dibattito sempre così appassionante sul sistema carcerario e sui livelli di sicurezza, si è omesso di sottolineare il fatto che nei primi due anni di questa legislatura

ai trattamenti penitenziari, sia necessario registrare questi dati e rilevare - come ha fatto il senatore Pedica, che con tanta forza

Dico questo perché evidentemente il trattamento dei detenuti è un problema serio all'interno del nostro Paese.

è materialmente impossibile che ci possano essere condanne che devono essere eseguite in carcere; semmai, si tratta di misure pre-cautelari eseguite

dopo l'arresto in flagranza e la convalida dell'arresto, queste persone sono espulse dal territorio nazionale e, nella stragrande maggioranza dei casi, non vi è l'accompagnamento coattivo. La violazione di questi ordini

di spaccio di sostanze stupefacenti l'80-90 per cento di questi traffici sia commesso da persone extracomunitarie irregolarmente presenti sul territorio nazionale. Signor Presidente,

giuridica. Se la legislatura rimarrà in piedi, occorrerà trovare i fondi e sostenere un provvedimento che riordini le carriere del personale della polizia penitenziaria perché, contrariamente al personale dei direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, il Corpo della Polizia penitenziaria è stato sempre escluso da provvedimenti di intervento. Credo anche

che si sacrifica. Nonostante sia al di sotto dell'organico di oltre 5.000 unità, il Corpo di polizia penitenziaria, con sacrifici individuali, è riuscito a gestire la situazione carceraria. Per questo,

Non è un provvedimento svuota carceri, né un provvedimento, caro senatore D'Ambrosio, simile ad un indulto.

norme, con previsione di sanzioni penali, rispetto a comportamenti illeciti,

Che cosa dovevamo fare? Dovevamo garantire che la detenzione domiciliare fosse una effettiva misura alternativa alla carcerazione. Perché vi fosse l'effettività della misura, era necessario innalzare la innalzare la pena per l'evasione a livelli tali da non rendere in alcun modo appetibile l'evasione dalla detenzione domiciliare, garantendo, attraverso l'aggravante specifica per eventuali reati commessi in quel periodo, un ulteriore inasprimento della pena. Questa è la valutazione complessiva che tutti dobbiamo fare.

Abbiamo già perso molto tempo e qualcuno ha ricordato che il provvedimento è stato approvato dalla Camera nel mese di luglio. Ma i tempi nel nostro Paese sono tali che abbiamo dovuto aspettare un ulteriore periodo per arrivare a questa soluzione.

come i cittadini percepiscono la vita carceraria nel carcere nel nostro Paese e su come valutano l'operato della Polizia penitenziaria. Si è trattato di un sondaggio disposto

non determinino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e nel presupposto, in relazione all'articolo 4 nella parte relativa alle assunzioni di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che vi sia il pieno rispetto dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. In relazione agli emendamenti, il parere è di nulla osta sugli emendamenti 4.1 e 4.100 nel medesimo presupposto riferito al testo. Esprime quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100, 1.200, 1.0.1

senatore Mazzatorta

a quei professori televisivi che usano tutti i mezzi per pubblicizzare i loro libri. Questa è la differenza tra chi lavora e chi chiacchiera. *(Applausi

mi accingo a trattare ho solo l'onore di illustralo, giacché rappresenta per intero la Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale, in tutte le sue componenti politiche, ma anche

Ci affidiamo al Governo e alla sensibilità dell'Aula per raccontare quello che abbiamo cercato di raccontare in ogni modo come Commissione, anche intervenendo sui *media* nazionali. Mi riferisco a un calvario che non è conosciuto

Noi abbiamo incontrato la dimenticanza totale della dignità umana; abbiamo incontrato uomini chiusi in luoghi non solo dove nessuno di noi - questo è chiaro - avrebbe desiderato essere ma dove non avremmo neanche pensato nel nostro ruolo istituzionale, anche ove fossimo stati semplici amministratori,

In quei sei ospedali psichiatrici giudiziari d'Italia noi abbiamo raccolto e nascosto sotto il più grosso dei tappeti la peggiore polvere immaginabile. Ripeto: la peggiore polvere immaginabile.

abbiamo incontrato persone che soffrono ancora di più, persone che non hanno più la speranza di tornare alla vita civile e ce lo hanno detto: «Noi non speriamo più», non perché stanno meglio lì, anzi vorrebbero ritornare, ma questo è un pensiero che nemmeno passa loro per la testa. Quante volte hanno incontrato il giudice di sorveglianza, quante volte hanno incontrato il medico, che ha finto - lo dico da medico - di realizzare programmi? Lì dentro, infatti, non si possono realizzare programmi di riabilitazione. Abbiamo visto film sulla legge Basaglia, ma dove è finita?

avrete letto dai giornali quando mi sono permesso di raccontare che costoro per rinfrescare l'acqua usavano il vano di un cesso: lì mettevano la bottiglia, perché era l'unico modo in cui potevano rinfrescare quello che, in una dura estate, in una stanza di carcere dove ci sono fino a dieci persone, potevano bere di fresco. Queste sono realtà, le raccontiamo a prescindere dalla parte politica; ci siamo sentiti onorati di firmare tutti insieme questo ordine del giorno, signor Sottosegretario, ma per noi occorre una sveglia particolare,

ma voglio pensare che sia anche un gesto importante. Anche oggi, convocando i rappresentanti degli assessori regionali alla sanità, abbiamo chiesto con loro non un patto

quante cooperative siamo tutti noi parlamentari interessati a seguire perché si dedichino a questi particolari servizi? Quante raccomandazioni per far sì che i contratti si rinnovino, che ci siano delle deroghe e che qualcosa vada avanti?

Vergogniamoci di sognarlo, di immaginarlo, vergogniamoci di una civiltà che rubiamo a questo Stato, ove quelle immagini venissero realmente rese pubbliche. Non si può andare in bagno davanti a tante persone: ebbene, lì vanno in bagno davanti a tante persone, non è concessa loro nemmeno quella dignità minima ed umana

Io so di essere legislatore, di aver avuto compiti e ruoli amministrativi, oltre che professionali, ma di fronte ad uno specchio che mi rimanda un'immagine così vergognosa,

per questa Aula, che vuole rappresentare con la stessa dignità quelle persone come tutte le altre che ha sempre rappresentato, sarebbe come un dono di Natale, l'inizio di un percorso diverso, di una sensibilità che accresce la dignità dello Stato e delle persone. *(Vivi applausi.

ci sono soldi disponibili per il recupero di questi pazienti che non vengono messi a disposizione per progetti territoriali. Bisogna che ci siano azioni concrete perché queste situazioni di vergogna nel Paese vengano superate. Sono poche cose, già stabilite. Basta attivarsi. Il Parlamento c'è. Chiediamo che anche il Governo, con coerenza, finalmente, faccia qualcosa per superare questa vergogna.

comporterebbe una serie di condizioni, precisazioni ed altro che non è il caso di valutare in questo momento. Quindi, una formulazione di questo tipo può andare bene.

del malfunzionamento del nostro sistema carcerario, del personale di Polizia penitenziaria. In generale, è quindi il problema che ha a che fare con le forze di polizia che, a vario titolo, garantiscono la sicurezza nel Paese. siamo almeno altrettanto contenti dell'avvenuta cattura di un pericolosissimo latitante e del successo ulteriore dell'attività investigativa delle forze dell'ordine e della magistratura. Nessuno che abbia un minimo di nozione di come funzionano queste cose potrebbe pensare che il merito di specifici atti di indagine, risultati investigativi, di specifiche catture di latitanti sia dell'autorità politica. su questi temi, più che su altri vi è una demagogia che andrebbe evitata. Congratulazioni quindi alla magistratura e alle forze dell'ordine - e basta - per il notevole successo conseguito.

con il precedente ordine del giorno illustrato dalla collega Della Monica, relativo alla necessità di un'integrazione complessiva del personale che opera nelle carceri. Quindi, parliamo di agenti di polizia penitenziaria, come prevede il testo di legge, educatori, come prevede l'ordine del giorno di cui abbiamo parlato prima, ma anche, inevitabilmente, di funzionari. Il meccanismo complessivo entra in sofferenza se non sono garantite tutte le parti dell'ingranaggio e in particolare non è possibile di nuove strutture penitenziarie, che pure esistono come edifici e come strutture fisiche, se, oltre alla polizia penitenziaria, intesa come agenti, come agenti, e agli educatori non vengono assunti in numero congruo e proporzionale ufficiali di Polizia penitenziaria, ed in particolare vice commissari. L'ordine del giorno G4.104 fa riferimento alla necessità di assunzione di vice commissari di Polizia penitenziaria, e ricorda come esista già un serbatoio di personale dal quale si può attingere, essendovi degli idonei di concorso che non sono stati dichiarati vincitori. Essi potrebbero essere assunti, quindi, in via straordinaria, con scorrimento della relativa graduatoria fino al numero ritenuto congruo in proporzione al numero di agenti di Polizia penitenziaria che si dovessero assumere. In questo senso, quindi,

G4.100 ed anche per rendere un po' di giustizia: anche in questi casi si vuole usare una punta di veleno. Io direi grazie ai magistrati, grazie alla polizia, ma grazie anche ad un'azione di governo che forse non ha mai avuto uguali fino ad oggi cosa che è interesse di tutti, crediamo. Il problema è che oggi ci sono pochi latitanti, non ce ne sono più, per cui per la polizia sarà sempre più difficile. Quello che vorremmo, poi, con questo ordine del giorno è di far funzionare al meglio gli istituti di pena, perché purtroppo sappiamo che con i trasferimenti si rischia di mettere a concorso dei posti e poi vedere vanificato o sguarnito un istituto perché, giustamente, tanti agenti hanno piacere a rientrare il più vicino possibile alle proprie abitazioni. Noi vorremmo un minimo di rigore, pensando all'interesse generale e al funzionamento della giustizia, per cui, una volta esperiti i bandi e assunti

È altrettanto sconveniente, oltre che inopportuno, che nessuno spenda mezza parola sul fatto che si consente ancora oggi sulle televisioni pubbliche, senza alcun tipo di contraddittorio, ad un qualsiasi giornalista che si improvvisa conduttore di sparare... sparare effettivamente delle sciocchezze ignobili: non tanto perché toccano il nostro partito, ma perché non hanno nessun peso, nessuna portata, nessuna validità, nessuna attinenza con la realtà. E non c'è nessuno che dica: possiamo anche pagare delle persone, ma nella televisione pubblica si diano notizie che siano notizie e che non siano pensieri. Anche noi abbiamo a cura e a cuore la condanna e la repressione della criminalità, ma non lo facciamo con questi slogan televisivi.

e siamo sodali con il ministro Maroni per la sua fatica: ce lo immaginiamo che scorre in armi campagne, contrade e città alla ricerca di quei latitanti che inutilmente i poliziotti cercavano da anni di catturare. È chiaro che questa enorme fatica nel ricercare i latitanti che la polizia e i carabinieri non riuscivano a catturare lo ha distratto dalle frequentazioni di qualche suo compagno di partito con gli 'ndranghetisti.

Continuate pure ad ululare, non mi impressiona il vostro ululato, anche se non siamo in cima alle montagne.

Scusate, sto parlando di un consigliere regionale che è stato fotografato insieme a un 'ndranghetista, tutto qui. Non è vero? È un falso fotografico?

Continuare il suo intervento, per esempio. LI GOTTI *(IdV)*. Mi voglio assicurare, Presidente, e lei me lo deve garantire, che nel verbale che poi verrà stampato ci sarà scritto "ululati". Lei interverrà sul processo verbale. Sono sicura che gli stenografi prenderanno sicuramente nota. Lei poi ha tutto il diritto di intervenire sul processo verbale, come sa. LI

ed era una delle parti di questo ordine del giorno, è che noi abbiamo pagato 200 miliardi di

si spendano 111 milioni di euro, ossia 200 miliardi di vecchie lire, per un braccialetto elettronico?

Quando pensiamo a questo dato, poi siamo costretti amaramente a raccogliere il dato contenuto nella legge di stabilità, che sottrae per il 2011 all'amministrazione penitenziaria 75,4 milioni di euro. Ossia, per il 2011, le già scarse risorse, già ridotte negli anni precedenti, vengono ulteriormente ridotte di 75,4 milioni di euro. Non vi indigna aver speso 200 miliardi di vecchie lire per un braccialetto elettronico e poi dover tagliare le risorse? Stiamo parlando di questi problemi. Negli interventi di molti colleghi è stata denunziata la gravissima sofferenza nel carcere che riguarda i detenuti e il personale della Polizia penitenziaria e quello amministrativo e, invece, i soldi li stiamo sprecando. Ci sono istituti carcerari

dopo due anni non è successo niente. Poi, sottosegretario Caliendo, è vero che il Ministero della giustizia non ha fatto sondaggi, però il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,

Obiettivamente, non vi sembra un po' ridicolo? Questi sono i contenuti del mio ordine del giorno.

favorevole a condizione che nella parte dispositiva, dopo le parole «impegna il Governo», sia scritto: «a valutare la possibilità di destinare gli agenti» e

Vorrei ricordare che soltanto con l'ausilio delle forze di opposizione e della maggioranza siamo riusciti a scrivere l'articolo 2 del disegno di legge sulla sicurezza,

procedere all'assunzione straordinaria di questo personale risultato idoneo, ma che non può essere probabilmente catalogato come "agenti".

alle Camere in merito al provvedimento, e chiede un impegno al Governo per definire una sorta di anagrafe degli istituti penitenziari,

aggiornato ogni sei mesi, accessibile, in forme digitali libere e aperte, da parte di chiunque ne abbia interesse attraverso il sito web del Ministero della giustizia, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento e fatte salve restrizioni dovute a comprovate ragioni

di boss mafiosi come Francesco Mannoia, Gaspare Mutolo, Totuccio Contorno, Giovanni Brusca, detto «lo scannacristiani» per la ferocia del suo agire criminale,

o in parte potrebbero non essere condivisibili. Quindi, nelle linee generali, andrebbe tenuto conto che in situazioni come quelle di grave allarme sociale si possa

utilizzare la memoria non in modo selettivo. Ricordo che in quest'Aula non vi è stata l'unanimità per l'articolo 2 del pacchetto sicurezza, perché molti senatori - non solo la senatrice Poretti ed io

è proprio dei giorni scorsi la costituzione, ad opera del nostro capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di un gruppo di lavoro con il precipuo compito di elaborare proposte di riorganizzazione dei circuiti detentivi e di possibili interventi normativi finalizzati a ridurre il sovraffollamento carcerario". Trascorsi due anni, il provvedimento è questo. Dei circuiti carcerari detentivi da riorganizzare non si è saputo più nulla; degli interventi normativi non si è saputo più nulla, eppure il problema esiste da anni esiste da anni e oggi viene risolto con una norma che si dice dice debba durare fino al 31 dicembre 2013, ossia in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario. Completa attuazione: noi non sappiamo nulla neanche dell'inizio dell'attuazione di questo piano straordinario. Allora riteniamo che le promesse fatte dal Governo, gli impegni assunti dal Governo non siano stati per nulla rispettati. Ora ci viene offerto questo provvedimento che sappiamo benissimo essere inidoneo a risolvere il problema, che è grave. Ricordavo poc'anzi che la scopertura degli agenti di Polizia penitenziaria ammonta a 6.000 unità e che il prossimo pensionamento vedrà aumentare questo numero di scoperture di altre 2.400 unità. A fronte di questo, si prevedono assunzioni forse, per 1.600 unità. Non basta la solidarietà, che pure è dovuta, a coloro che svolgono il lavoro difficilissimo della custodia di chi è in carcere: non basta la solidarietà, non basta ringraziarli, ci vogliono provvedimenti ed è impensabile che dopo anni e anni ancora non si riesca a risolvere questo problema. motivi, il nostro voto si limiterà all'astensione, come segnale di attenzione verso un problema che esiste, ma anche come segnale di denunzia per un problema che non vediamo essere risolto con impegni seri e realizzabili in termini certi. Mi deve consentire, signora Presidente, visto che sono state enunciate alcune affermazioni sul mio conto, di dire che è assolutamente vero che io nel 1980, richiesto da Giovanni Falcone, assunsi la difesa di collaboratori di giustizia che nessuno voleva difendere. L'ho fatto per senso dello Stato e per rispetto della mia dignità e della deontologia professionale.

E l'ho continuato a farlo sino a qualche anno fa, pur se, ancora nel 2007, come risulta da documenti ufficiali, Totò Riina in carcere commissionava al clan Misso il compito di eliminarmi con un attentato dinamitardo. il 26 novembre 2007, tanto è vero che lo Stato si fece cura di garantirmi - non da me richiesta - una forma di protezione. Queste sono scelte difficili, che si compiono onorando il dovere dell'avvocato e per senso dello Stato. È difficile comprenderlo, ma io sono orgoglioso della mia scelta.

Signora Presidente, mi consenta prima di tutto di congratularmi con la magistratura e con il Ministero dell'interno (e con Ministero dell'interno intendo il ministro Maroni le forze di polizia) per i recenti successi ottenuti in tema di mafia e di lotta alla criminalità organizzata. non parlo di polizia e magistratura perché, dato il mio precedente lavoro, sembrerebbe un discorso settario, ma devo congratularmi con il Ministro perché, nonostante questo Governo abbia effettuato tagli macroscopici alle forze dell'ordine, egli è riuscito a tenere alto il morale

la guerra contro la mafia si vince in un altro modo, e nessun Governo si è mai interessato a vincere la guerra, perché la guerra contro la mafia si vince con il lavoro e con

Non capisco poi perché noi ci siamo soffermati a parlare di questo, quando il provvedimento in esame recita tutt'altra cosa. Nell'annunciare il voto di astensione del mio Gruppo, nella speranza che in tema di carceri non ci sia più uno stato di emergenza che ci costringa a questo, e ritenendo di fare cosa gradita a tutti i colleghi, consegnerò il testo integrale del mio intervento.

Presidente, noi voteremo a favore di questo provvedimento come misura emergenziale e temporanea, vista la sua scadenza nel 2013, 2013, e voteremo anche per i quattro punti che sono ben chiari nel testo del provvedimento: l'esclusione per i reati di maggiore allarme sociale; il fatto che non vi sia nessun automatismo, perché l'autorità giudiziaria ha un ampio margine di valutazione nella concessione della detenzione domiciliare;

la previsione di una nuova circostanza aggravante (nel senso che, se il detenuto si allontana dell'abitazione e commette un reato, ci sarà un aggravamento della pena); infine, l'adeguamento dell'organico della polizia penitenziaria, che permetterà di fronteggiare la situazione emergenziale. Per questi motivi, noi voteremo a favore del provvedimento.

per la brillante attività investigativa che ha condotto alla cattura del *boss* latitante Antonio Iovine. I complimenti sono da rivolgere alle forze dell'ordine, alla magistratura, nonché al Parlamento che ha varato norme efficaci nella lotta alla criminalità. Al contempo va fortemente respinta e condannata l'intimidazione che anche da quest'Aula è partita nei confronti di Roberto Saviano, che si è solo limitato a parlare di fatti. Signori della maggioranza e del Governo, se la verità vi fa male o vi dà fastidio, oppure se avete la coda di paglia, sono affari vostri, ma non cercate di attaccare la libertà di stampa e di espressione. Venendo al disegno di legge, esso si inserisce nel quadro della politica di deflazione carceraria annunciata dal Governo in occasione dell'adozione del cosiddetto piano carceri. L'obiettivo dichiarato dell'intervento legislativo è quello di arginare il sovraffollamento carcerario senza sospendere l'esecuzione della pena attraverso la forma dell'esecuzione domestica. L'obiettivo governativo, però, non è stato purtroppo affatto raggiunto. Il testo in esame ripropone una specie di detenzione domiciliare che presta il fianco a critiche di coerenza sistematica, che pone forti dubbi da un punto di vista anche processuale e che - soprattutto - non risolve il problema emergenziale e i problemi fortissimi di illegalità all'interno delle carceri, dove continuano a verificarsi morti e suicidi. Come Partito Democratico noi eravamo d'accordo, già nell'ambito dei lavori svolti presso la Camera dei deputati, rispetto alla scelta di affrontare convintamente e urgentemente questo disegno di legge, tanto è vero che alla Camera si è votato favorevolmente e che anche in questa sede abbiamo ritirato i nostri emendamenti. Questa è stata una sorta di apertura di credito nei confronti delle promesse fatte dal Governo. Però abbiamo dovuto osservare che dal luglio del 2010 (da quando c'è stato il voto alla Camera) il Governo non ha fatto assolutamente nulla: il piano carceri continua a rimanere fermo, sulle misure alternative al carcere non è entrato in vigore assolutamente nulla e sulla depenalizzazione nulla si è detto.

quelli del sovraffollamento, della carenza del personale di sorveglianza e dell'insufficienza del personale in grado di fornire assistenza sociale e psicologica in carcere. Abbiamo presentato dei disegni di legge volti a supportare queste misure; abbiamo proposto l'adozione di un patto per il reinserimento e la sicurezza sociale; abbiamo proposto di adeguare le piante organiche del personale della Polizia penitenziaria; abbiamo chiesto la revisione delle norme sulla custodia precautelare e sulla custodia cautelare in carcere, limitandola a criteri più stringenti per il suo utilizzo. Abbiamo anche proposto l'istituzione di un garante nazionale delle persone private della libertà personale, indipendente e articolato localmente, che si possa coordinare con tutti i garanti comunali e provinciali esistenti. C'è stata una risposta praticamente nulla da parte del Governo e della maggioranza. L'unico aspetto positivo che ritroviamo in questo disegno di legge ci viene fornito dall'articolo 4, riguardante le assunzioni del personale della Polizia penitenziaria. Però, anche in questo caso, ancora una volta, c'è un rinvio che viene fatto dal Governo alla legge di stabilità. C'è quasi una sorta di presa in giro. Come Partito Democratico, preso atto della situazione di emergenza ricordata da tutti in quest'Aula, avevamo operato, come dicevo, questa sorta di apertura di credito a favore della politica carceraria del Governo enunciata più volte ai *mass media,* e anche in quest'Aula. Parlavo del voto favorevole alla Camera e del nostro comportamento in Commissione e in quest'Aula contro l'allungamento dei tempi e sostenendo le esigenze dell'urgenza. Ma ancora una volta il Governo, e in particolare il Ministro della giustizia, ha perso tempo e ci ha fortemente deluso, perché ancora una volta, in materia di giustizia, ci sono state solo parole, parole e parole. Non vogliamo essere presi in giro: non prendete in giro, signori del Governo, gli operatori del sistema carcerario; non prendete in giro gli italiani. Come Partito Democratico, abbiamo avanzato proposte concrete e precise: aspettiamo ora che il Governo e il Ministro della giustizia rispettino gli impegni presi. Per senso di responsabilità, civica e politica, non abbiamo voluto bloccare questo provvedimento né rallentarne l'*iter:* provvedimento che non ci entusiasma, ma che apre delle possibilità. Vedremo se con la legge di stabilità prossima ventura il Governo coprirà i buchi finanziari e le perplessità che scaturiscono da questo disegno di legge. Per il momento, essendo per tutti evidente la necessità di ampliare il numero degli addetti professionali al sistema carcerario nel loro insieme, ci limitiamo all'astensione, segno della nostra concreta volontà di riportare legalità e funzionalità all'interno del mondo penitenziario, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dalla nostra Costituzione.

Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, credo che sia innanzitutto, non opportuno, ma doveroso ringraziare le forze dell'ordine

...applicando gli stessi principi che l'opposizione ha applicato non più tardi di tre o quattro giorni fa quando, a seguito del crollo di uno delle migliaia e migliaia di monumenti che danno prestigio alla nostra Italia, sono venuti qua a chiedere al ministro Bondi di dimettersi: ma come, quando le cose vanno male la colpa è del Ministro e quando le cose vanno bene non è merito del Ministro? Signori senatori, questo provvedimento certo non risolve i problemi delle carceri non risolve i problemi delle carceri italiane, ma è qualcosa che sicuramente avrà degli effetti positivi. È un provvedimento studiato con molta attenzione, perché bisogna considerare che non è che quando manca un anno alla fine della pena immediatamente il detenuto esca dal carcere; non è così: quando manca un anno al termine della pena, viene incaricato il giudice di sorveglianza di valutare se quel detenuto ha la possibilità di essere rimesso in libertà,

aggiunta all'articolo 61, comma 11, del codice penale per chi commette reati essendo stato assegnato agli arresti domiciliari. È sicuramente una norma

siano sotto sorveglianza e, se violeranno le norme che consentono di essere messi agli arresti domiciliari, abbiano delle pene assai gravi. Questa è la prima parte del disegno di legge. La seconda parte del disegno di legge è quella che fa qualcosa di positivo per coloro che nelle carceri lavorano, e che ci lavorano con grandi sacrifici; chi come me fa l'avvocato penalista e quindi ha occasioni frequenti di andare in carcere se ne rende perfettamente conto: conto: si impegnano in un lavoro difficile, nel quale bisogna contemperare l'esigenza di far rispettare la disciplina che deve governare

solo una battuta, signora Presidente: l'esercizio della verità non è mai una cosa positiva, sia quando riguarda i Ministri, sia quando riguarda i magistrati, sia quando riguarda le forze dell'ordine.

Migliaia di persone quotidianamente subiscono una vera e propria tortura per il modo con cui sono ristrette negli istituti di pena italiani. Il Parlamento non ha saputo dare una risposta, anzi si è adoperato per peggiorare la minima proposta di riduzione del danno che si infligge quotidianamente fatta dal Governo. Occorrerà quindi portare la questione a livello sociale, perché si tratta di un problema sociale, e di ampliare mobilitazioni non violente che vogliano riportare al centro - questo lo dico in particolare ai colleghi del Gruppo del Partito Democratico - il rispetto quotidiano della Costituzione, indipendentemente da chi poi ne subisca le conseguenze. È il caso di unirsi all'iniziativa non violenta che Marco Pannella porta avanti da 45 giorni anche per vedere la nostra

finestra") ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

un minuto per ravvivare l'interesse dei colleghi su questo provvedimento, che adotta uno schema consolidato internazionalmente per evitare la doppia imposizione e che per l'Italia riguarda le imposte IRPEF, IRPEG

Governo, invito il senatore Segretario a dare lettura del parere della 5a Commissione «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto della natura meramente eventuale e non previamente quantificabile degli effetti di gettito. Il parere è altresì reso con la seguente osservazione: la Commissione, pur preso atto degli elementi forniti dal Governo circa la compatibilità della riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170, in materia di desertificazione, con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente, evidenzia, secondo quanto già rilevato con riferimento ad altri provvedimenti di ratifica di accordi internazionali, che la modalità di copertura impiegata nel provvedimento non debba essere reiterata per la copertura di futuri accordi internazionali ed invita il Ministero dell'economia e delle finanze ad individuare preventivamente modalità di copertura alternative più conformi alla legge n. 196 del 2009 per altri provvedimenti di ratifica, recanti identica copertura, già presentati alle Camere e non ancora discussi».

DISEGNO DI LEGGE Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta La relazione è stata già stampata e distribuita.

invito il senatore Segretario a dare lettura del parere della 5a Commissione che sia inserito un articolo recante: "Clausola di monitoraggio" con le seguenti parole:

Brasile nei vari campi di sicurezza, difesa, supporti logistici, formazione militare, esperienze acquisite in operazioni umanitarie ed altre. ha durata illimitata e non comporta oneri a carico dello Stato, come spiegato nella relazione tecnica. Pertanto, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di

indubbiamente il Brasile è quello più vicino all'Italia per ragioni storiche e culturali, e quindi tutto ciò che è investimento sul futuro di quel Paese, anche in un campo delicato come quello della difesa, non può che essere guardato positivamente.

intervengo a seguito dell'annuncio fatto stamane dal collega Perduca, (che non vedo in Aula ma che leggerà il Resoconto), di un'interrogazione circa le manifestazioni di Brescia e Milano - la mia città - di cittadini stranieri che attendono il rinnovo del permesso di soggiorno. Lunedì scorso io ero presente al presidio organizzato presso il consolato egiziano a Milano e all'assemblea sotto la torre di via Imbonati, dove da alcuni giorni molti lavoratori protestano. Purtroppo, si sta verificando quanto avevamo già previsto a suo tempo quando è stato approvato il cosiddetto pacchetto sicurezza ed oggi è davvero alto il rischio che la situazione possa esplodere in tutta Italia. Preciso al collega Perduca che non possiamo sottoscrivere un'interrogazione che si basi sul congelamento dell'espulsione dei lavoratori immigrati in quanto, come Italia dei Valori, siamo rispettosi delle leggi, anche quando non ci piacciono: questo è il principio di legalità. È necessario invece intervenire per modificare l'assurda legislazione vigente, che prevede il reato di clandestinità per chi rimane nel nostro Paese senza lavoro.

volto a modificare il testo unico che disciplina l'immigrazione. Il nostro emendamento prevede, sotto il profilo normativo, la proroga del permesso di soggiorno per altri 12 mesi per coloro che rimangono privi di occupazione per cause indipendenti dalla loro responsabilità. Riteniamo che questo emendamento possa essere risolutivo, normativamente, della situazione che purtroppo si è venuta a creare.

I lavoratori della Eaton di Massa Carrara, durante un corteo sindacale, sono stati inopinatamente e brutalmente caricati dalle forze dell'ordine. La dinamica è presto raccontata. I lavoratori in corteo, in modo assolutamente pacifico, escono dalla fabbrica per andare incontro al prefetto, che torna da Roma con notizie sulla loro vertenza, su cui poi dirò alcune cose. A 100 metri dal casello dell'autostrada, senza ragione alcuna e senza alcun preavviso, e soprattutto senza che i lavoratori avessero minimamente come obiettivo di occupare l'autostrada, è partita una brutale carica delle forze dell'ordine; i lavoratori, con le mani alzate, sono stati caricati con brutalità. Due dirigenti sindacali, Alessio Castelli e Gioacchino Pitanti, sono ricoverati in ospedale. Innanzi tutto, voglio inviare a loro, interpretando, ne sono certo, il pensiero dei colleghi, i più calorosi auguri di pronta guarigione. Conosco quei lavoratori e quei dirigenti sindacali e sono stato con loro più volte in queste settimane: sono persone che stimo moltissimo; sono lavoratori, non ultrà da stadio. Sono 350 persone che da due anni sono in cassa integrazione, che, vi assicuro, non è una bella condizione, per giunta senza certezza per il loro futuro. Sono 350 lavoratori costretti da due mesi ad occupare la loro fabbrica, e questo perché la multinazionale Eaton, come sempre più spesso accade per le aziende a capitale estero, con totale disinteresse per il territorio che l'ha ospitata per anni, dal quale ha tratto importanti benefici, decide di chiudere quel L'unica certezza per quei lavoratori è la scadenza del 14 dicembre, data nella quale cessa la cassa integrazione e cessa quindi ogni forma di reddito. Per questo, quei lavoratori hanno aspettato l'incontro di ieri al Ministero dello sviluppo economico con un carico alto, molto alto, di speranza, come l'ultima possibilità per ottenere un periodo di cassa integrazione in deroga per il tempo strettamente necessario affinché l'impegno totale e importantissimo delle istituzioni locali a tutti i livelli per trovare progetti credibili di reindustrializzazione potesse concretizzarsi positivamente. Vede, signora Presidente, quei lavoratori non vogliono assistenza, vogliono lavorare, guadagnarsi lo stipendio con il loro lavoro. Bene, e cosa succede nell'incontro di ieri? Che questa multinazionale, assolutamente indifferente alla situazione sociale che essa stessa ha prodotto con la decisione di chiudere quel sito produttivo, si dichiara indisponibile a tutto, cosa questa che fa anche alterare gli stessi membri Questi sono i fatti. Le chiedo, signora Presidente, di farsi interprete presso il Ministro dell'interno affinché venga in Aula o in Commissione a riferire delle responsabilità gravissime che si sono rese evidenti

Signora Presidente, vorrei esprimere la solidarietà del nostro Gruppo, e mia personale, ai lavoratori della Eaton ed a questa battaglia importante che il mondo del lavoro affronta ogni giorno sul terreno della competitività internazionale. dire al collega Passoni, che è un rappresentante sindacale, che credo sia del tutto fuori luogo sostenere che vi siano state brutalità, cariche e interventi inopinati. Vorrei, quindi, che questo dibattito fosse sereno, in un Paese in cui il controllo sulla legalità e l'uso della forza è rimesso alla competente autorità giudiziaria. Non vorrei, in altre parole, che

debba essere sottolineato un elemento importante: lo sforzo del Governo, che sta cercando, in questi anni di crisi internazionale, di trovare gli ombrelli e gli ammortizzatori sociali necessari per far fronte a questa crisi e alle esigenze del mondo del lavoro. Non voglio neppure dimenticare

La seduta è tolta